La seduta è aperta

il più grave difetto di un politico e anche di chi ci governa abitualmente è quello di non sapere guardare in faccia la realtà: si dovrebbe governare quello che esiste e non quello che si vorrebbe esistesse. Anche a noi piacerebbe che nel mondo non ci fossero guerre, carestie e dittature, che spingono milioni di persone a scappare dalle loro case e dalle loro Nazioni. Ci piacerebbe anche che le ondate migratorie non fossero in mano ad esseri spregevoli, che lucrano sulla sopravvivenza e sul dramma degli individui, che uccidono e lasciano morire e che spesso, guarda caso, sono legate al terrorismo. Ci piacerebbe anche che la parte ricca del mondo potesse accogliere tutti con dignità, fornire loro alloggi, cibo, lavoro e conoscenze, senza richiuderli in *lager*. Purtroppo la realtà è completamente diversa, caro Vice Ministro: che il Governo ne prenda atto

baraccopoli nate intorno alla tragedia umana di questi migranti, nei campi di raccolta dei pomodori e guardate finalmente in faccia la realtà. «In tema di immigrazione è tempo di prendere atto che le condizioni intorno a noi sono profondamente mutate. Non definiamola più emergenza: oggi siamo nel pieno di una dolorosa e costante problematica da gestire» E ancora: «Oggi l'immigrazione non è un cerino da passare di mano in mano. È una questione gigantesca che chiede un radicale cambio di passo a livello nazionale. O daremo sostanza a questo cambio di passo o finiranno per prevalere egoismi e paure, che porteranno altri milioni di voti ai populisti di ogni genere». Queste parole non le abbiamo dette noi, ma le ha scritte Sala, sindaco della più importante città italiana, del Partito Democratico. Anche il Presidente della Regione Sardegna, Pigliaru, che mi sembra essere vicino a SEL, ha dovuto scrivere l'altro giorno al ministro Alfano per evitare che una nave norvegese sbarcasse sulle coste sarde e ha chiesto e imposto che venisse dirottata a Palermo: non ha accettato che altre mille persone arrivassero in Sardegna. Nell'ultima settimana sono arrivati 11.000 profughi; complessivamente sono 157.000 contro i 170.000 di tutto il 2014. Tra di loro ci possono essere terroristi (nessuno lo sa), potranno diventare manodopera a basso costo per la criminalità comune e organizzata; quante donne saranno costrette a prostituirsi? Quanti ragazzi saranno obbligati a spacciare e a rubare?

anzi è il Governo che non ha consentito - di entrare nella fase 2, quella finale, cioè di entrare nelle acque territoriali libiche per distruggere là le barche che non devono partire cariche di profughi. Sappiamo benissimo dove sono le basi e dove sono i gommoni. Tutti gli altri Paesi sono più attivi di noi, come hanno dimostrato gli americani bombardando Sabrata e uccidendo in un solo bombardamento più di 50 terroristi. Si sta muovendo anche il generale Aftar,

caro Sottosegretario, sembra essere l'unica che conoscete, come nel caso del documento dell'UNESCO.

e il mondo alla rovescia nel quale, purtroppo per l'Italia, ancora credete, non esiste: la realtà vi si ribalterà addosso e vi schiaccerà. Probabilmente schiaccerà tutto il Paese e tutti noi.

colleghi, rappresentante del Governo, con i 12.000 sbarchi degli ultimi tre giorni abbiamo toccato ieri il numero di 153.450 arrivi solo nel 2016. Non solo c'è un aumento del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (peraltro, con gli arrivi di oggi supereremo il totale del 2015 e mancano ancora oltre due mesi per giungere alla fine dell'anno), ma viene anche superato il 2014, anno *record*, chiuso con 170.000 arrivi. Sottolineo che da quando c'è Renzi al Governo gli sbarchi in Italia sono quasi mezzo milione. Questo non dovrebbe succedere in un Paese serio che attua una politica di gestione degli immigrati basata su legalità e deterrenza. Succede invece nel nostro Paese che fa esattamente il contrario: non contrasta adeguatamente gli scafisti, legalizza la clandestinità e poi pratica l'assurda politica delle frontiere aperte e della riduzione dei controlli terrestri. Sottolineo un dato: dei circa 11.000 pachistani che nel 2016 hanno chiesto asilo, nessuno è entrato via mare ed è contabilizzato in quel numero dei 153.000; questo vuol dire che l'Europa paga a Erdogan fior di miliardi solo per fermare i siriani, ma non altre nazionalità. Inoltre è assurdo che questi pachistani entrino dalla Slovenia e dall'Austria, dove noi non pretendiamo l'applicazione della regola del Paese di primo approdo. Abbiamo un sistema di accoglienza al collasso, con oltre l'80 per cento dei presenti collocati in strutture temporanee, abitazioni private e alberghi. Siamo arrivati ieri a 166.921 migranti accolti. Questo perché c'è una lentezza nella valutazione delle domande d'asilo, perché sono poche le commissioni di valutazione, perché sono pochi gli operatori all'interno delle commissioni e di quei pochi che ci sono, pochi lavorano a tempo pieno; perché c'è una giustizia ordinaria che capovolge gli esiti di prima istanza e che persino riconosce la condizione di migrante economico, meritevole di protezione internazionale, sovvertendo i principi internazionali dell'asilo. quella stessa parte di magistratura politicizzata che indaga persino i nostri marinai della guardia costiera per non essere riusciti ad evitare il naufragio dei barconi. È un disastro perché accogliamo migranti che vengono dell'Africa subsahariana, dall'Africa centrale, cioè migranti economici, che sono clandestini. Stiamo parlando di nigeriani, di personalità del Gambia, del Mali, del Senegal, della Costa d'Avorio, dove le statistiche del Ministero dell'interno dicono che una percentuale inferiore al 5 per Lo scorso anno Padoan parlava di 3,3 miliardi di soldi spesi per l'accoglienza; quest'anno siamo ad oltre 4 miliardi. È una gestione disastrosa;

Il sistema di accoglienza, come ho detto prima, è al collasso; quasi 4 su 5 dei migranti e richiedenti asilo sono nelle strutture temporanee.

il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 142 del 2015, approvato dalla maggioranza in Commissione affari costituzionali, un richiedente asilo può essere iscritto all'anagrafe comunale e può richiedere anche la carte d'identità, con numerose incombenze a carico dei Comuni, soprattutto quando si verificano fenomeni di irreperibilità. PRESIDENTE. e denaro per i Comuni che devono affrontare in merito a questo aspetto. È per tale motivo che noi abbiamo presentato questa mozione impegna il Governo a modificare rapidamente questo decreto legislativo, che presenta buchi e criticità, come ha ammesso anche, stranamente, il prefetto Morcone la scorsa settimana in occasione dell'audizione del Comitato Schengen.

in termini economici e sociali sul nostro Paese. Questo lo denuncio.

«Come può uno scoglio arginare il mare», credo però che siamo di fronte ad un fenomeno talmente vasto ed epocale che non basteranno muri, reticolati, respingimenti Da qui dobbiamo partire. E forse il processo, invece che al Governo, andrebbe fatto all'Unione europea, che dietro l'usbergo di decine di regolamenti, di direttive e di agende ha poi sposato pragmaticamente la filosofia "dell'ognuno si faccia i fatti suoi". Di conseguenza,

sui ritardi, sulle carenze vistose dell'Unione europea per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. La risposta è stata tardiva e risale al maggio 2015, con l'agenda europea per la migrazione, che aveva degli obiettivi eccellenti: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, salvare le vite umane, rendere sicure le frontiere esterne, garantire l'attuazione del sistema europeo comune di asilo promuovendo su base sistematica l'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali, realizzare una nuova politica di migrazione locale. Ebbene, dopo oltre un anno dalla presentazione dell'agenda, il bilancio è fallimentare. A fronte di una serie di misure adottate per ridurre i flussi irregolari verso e all'interno dell'Europa e per proteggere le frontiere esterne europee, in particolare l'aumento delle capacità e delle risorse disponibili nel 2015 e 2016 per le operazioni Triton e Poseidon di Frontex, l'adozione dell'approccio *spot* e l'intesa con la Turchia del marzo 2016, l'Italia e la Grecia continuano ad essere l'unico approdo possibile, e rimangono gli unici Stati competenti all'esame delle domande di asilo, come previsto dal regolamento di Dublino. I numeri ridicoli dei meccanismi di ricollocamento e reinsediamento confermano il fallimento del tentativo di assicurare una maggiore e più equa condivisione della gestione dei flussi. si innesta un altro grande problema, quello che la migrazione non può essere lasciata fuori controllo. Esiste, infatti, un tasso ottimale di immigrazione, oltre il quale questo processo genera costi per tutti: per i Paesi d'arrivo e per gli stessi migranti. però, sono spietati. Un anno dopo il varo del progetto di ricollocamento tra gli Stati europei, il numero complessivo dei richiedenti asilo trasferiti dall'Italia verso altri Paesi è ancora fermo al 3 per cento dell'obiettivo, ovvero 1.196 persone su un totale previsto di 39.600. Dal 12 luglio al 27 settembre, 2242 persone si sono spostate dalla Grecia, e appena 353 dall'Italia. A fronte di questo, la proposta di riforma del regolamento di Dublino presentato dalla Commissione europea lo scorso 4 maggio pretende di rimediare all'evidente fallimento del sistema Dublino, mantenendo sostanzialmente invariata la gerarchia dei criteri Dublino. la nostra mozione è impegnata su questo: alzare la voce in Europa per modificare davvero il regolamento di Dublino. rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il Senato torna oggi ad affrontare il problema della crisi derivante dall'aumento esponenziale dell'afflusso di migranti in fuga dai propri Paesi d'origine, che, come sappiamo, trae origine dall'ormai cronica instabilità politica che caratterizza il bacino del Mediterraneo e l'Africa sahariana e subsahariana. I conflitti costanti hanno determinato una gravissima crisi umanitaria di enormi proporzioni, che ha riversato sulle coste dei Paesi di primo approdo (in particolare Grecia e Italia) un numero in continua crescita di profughi.

con l'ingresso di ulteriori 154.000 migranti. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati in Italia e Grecia è costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godrebbero comunque di un alto tasso di riconoscimento a livello di Unione. Mi permetto inoltre di ricordare che, secondo i dati Eurostat, nel 2015 i richiedenti protezione internazionale in Italia sono stati 83.540, mentre erano stati 64.625

simultaneamente: ricollocazione-reinsediamento; rimpatrio-reinserimento; cooperazione con i Paesi di origine e di transito. Tali principi sono stati recepiti in due decisioni del Consiglio del settembre 2015, che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, prevedendo, nel complesso, un totale di persone da ricollocare pari a 160.000 unità, di cui circa 39.600 dall'Italia. Tuttavia, il più recente sesto rapporto della Commissione europea del 28 settembre 2016 ha evidenziato un sostanziale fallimento di questo meccanismo di ricollocamento dei richiedenti asilo fra gli Stati membri, in quanto, dopo un anno circa, sono state ricollocate solamente 5.651 persone, delle quali 1.196

Alla base di tale fallimento vi è una molteplicità di fattori, quali il numero insufficiente e limitato di impegni formali da parte degli Stati membri assegnatari di quote dei migranti (Croazia, Ungheria e Slovacchia non hanno reso disponibili posti posti di ricollocazione), un uso scorretto delle preferenze da parte degli Stati membri, tempi talvolta lunghi di risposta alle richieste di ricollocazione e ostacoli inerenti ai controlli di sicurezza o, addirittura, rigetti del tutto ingiustificati. Vorrei in particolare stigmatizzare un fatto di particolare gravità, ossia la problematicità della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. L'arenarsi del piano di ricollocamento è solo uno dei preoccupanti aspetti riconducibili a un'inversione di tendenza, un cambiamento di orientamento, ravvisabile nei recenti atti di provenienza europea regolanti la gestione dei flussi migratori, dai quali emerge un complessivo indebolimento del diritto di asilo in Europa. Si va in effetti verso una precarizzazione della protezione internazionale in ambito europeo, con un ulteriore appesantimento degli obblighi previsti per i Paesi di primo approdo. L'atto che ho presentato intende fornire al Governo delle indicazioni per invertire questa tendenza, perché sono fermamente convinto che è possibile avere una migrazione diversa, basata sulla riduzione del numero di vittime, attraverso il attraverso il rafforzamento delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e la realizzazione dei cosiddetti corridoi umanitari; sulla lotta alla tratta, sulla possibilità per i migranti di effettuare giustificati movimenti secondari all'interno del territorio dell'Unione, nonché rendere più efficienti e concrete le procedure regolanti le domande di protezione internazionale. internazionale. Ma tutto questo è impossibile se l'Unione non prenderà un impegno concreto a mantenere saldi i principi alla base dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: solidarietà, rispetto per la vita umana e condivisione degli oneri.

a destra invece hanno urlato «respingiamoli tutti» e infatti abbiamo visto che erano legati a Mafia Capitale e gestivano i migranti che erano più redditizi della droga e della prostituzione. C'è una cosa che accomuna però destra e sinistra che è la decisione sugli interventi militari interventi militari italiani in giro per il mondo: vi sono stati l'Afghanistan, l'Iraq, la sconfitta della dittatura di Gheddafi; adesso abbiamo il caos in Siria, perché siamo finanziando gruppi islamici salafiti armandoli e spedendoli in Siria a combattere contro i siriani. siete ancora tutti d'accordo sul traffico di armi verso l'Arabia Saudita per combattere la popolazione civile dello Yemen. Ebbene, ciò che dovremo fare è innanzitutto mettere in relazione la politica estera La nostra politica estera sta determinando non soltanto migranti politici (quindi richiedenti asilo), ma anche nuovi tipi di migranti, ad esempio i migranti per fame, i migranti economici, e addirittura i migranti ambientali: milioni di profughi che si sommano ai profughi storicamente noti; persone che scappano dell'inquinamento delle multinazionali, anche italiane: ad esempio, l'ENI nel Delta del Niger; diamanti, coltan, monocolture nel Sahel e in altri luoghi dell'Africa. Questo stiamo facendo in giro per il mondo. Tutto questo ha dei costi enormi anche in Italia: l'accoglienza ci costa circa 100 milioni di euro ogni mese (1,2 miliardi l'anno). E gli sbarchi stanno aumentando: gli arrivi in Italia sono giunti a quota 160.000 - è già stato detto - e sono raddoppiati con Renzi, che ha questa favolosa tendenza a dichiarare che il numero diminuisce, quando invece raddoppia, anche in questo caso. Quelli che invece non aumentano sono i rientri: stiamo parlando di 5.000 persone circa su 160.000 arrivi cento). Come stiamo gestendo tale questione? Abbiamo una missione navale, EUNAVFOR Med, totalmente insufficiente e inadeguata, perché le morti nel Mediterraneo continuano ad esserci e sono aumentate. L'Unione europea ha dimenticato il Mediterraneo perché ha pensato di bloccare una rotta, quella balcanica, siglando con la Turchia un accordo scellerato e miliardario. c'è quello che non sta facendo. Tutti stiamo chiedendo e chiederemo questa mattina la riforma, il superamento del sistema Dublino III; ma i pacchetti proposti in Commissione europea a noi sembrano assolutamente non sufficienti e sono, di fatto, una non riforma. A margine di tutto questo, nonostante le audizioni fatte qui in Senato, per i nostri cittadini, per i Comuni che sono ai confini della nostra Italia, ma che sono anche i confini europei,

Chiediamo assolutamente una riforma che cancelli il principio dello Stato di primo approdo; chiediamo che sia attuata per tutti gli Stati membri una più equa ripartizione, quindi l'introduzione di quote di distribuzione dei migranti; la sospensione della missione EUNAVFOR Med; vogliamo che sia favorito un sistema di accoglienza diffuso dei migranti, che non vada a pesare solo su determinati Comuni italiani; che siano potenziate le commissioni di valutazione dei richiedenti asilo; che sia implementata la diffusione del sistema SPRAR, che sta funzionando, e che vengano intensificati i controlli e le forme di assistenza ai minori. Tutto questo in una gestione quanto più trasparente.

per il nostro Paese la questione meridionale. Essa, infatti, interseca le modalità di declinazione della convivenza umana, ridisegna i confini geografici e politici, oltrepassa barriere fisiche e culturali, accentua le differenze per poi annullare la diversità per ricordarci che siamo tutti cittadini del mondo. Nella partita dell'immigrazione si gioca la nostra stessa identità di cittadini e il senso vero che diamo alle parole: inclusione, integrazione, diritto ad avere diritti. La partita è a tutto campo, perché la sfida è nello stesso tempo a livello internazionale, nazionale e di prossimità, nei nostri territori. Per questo la nostra mozione è ambiziosa e impegna il Governo su una pluralità di fronti, a cominciare dall'Unione europea e oltre i suoi confini. Il tema dell'asilo, un diritto di asilo europeo, deve tornare al centro del dibattito europeo, rilanciando la necessità di abolire il regolamento Dublino III e le quote di redistribuzione dei richiedenti asilo, che non tengono conto dei legami familiari allargati, promuovendo l'apertura immediata di corridoi umanitari e permessi di soggiorno per coloro che scappano da persecuzioni e guerre; mettendo in campo iniziative per accelerare la regolarizzazione e fermare i respingimenti verso i Paesi di origine. Molti sono gli accordi con specifici Paesi, come la Turchia, che dovrebbero essere cambiati; intollerabili quelli con i Governi che non rispettano i diritti umani. Anche per questo chiediamo che l'accoglienza divenga presupposto dirimente per la partecipazione degli Stati all'Unione europea. Occorrono un piano nazionale di accoglienza, in grado di valorizzare l'impatto economico e sociale dei migranti; una legge organica sul diritto d'asilo e un monitoraggio costante della sua attuazione; il riordino delle forme di accoglienza, in sinergia con gli enti locali e le associazioni di volontariato, per arrivare alla chiusura definitiva dei centri di identificazione ed espulsione e delle macro-strutture come i CARA di Mineo e di Bari, dove sono state scritte pagine vergognose che - come Sinistra Italiana-SEL - abbiamo sempre denunciato. Io stesso a febbraio scorso ho presentato un'interrogazione sul CARA di Casale San Nicola a Roma. un'esperienza straordinaria di giovani immigrati che, per responsabilità di quattro facinorosi, fa arretrare lo Stato. Vergognoso! Il nostro obiettivo deve essere uno su tutti: il pieno inserimento degli immigrati nella collettività, attraverso formazione, lavoro, mediazione culturale, condizioni

umanamente, ha orrore della tratta degli esseri umani, della schiavitù, della violenza alle donne e delle stragi del mare e ne auspica la fine immediata. Per questo la nostra risposta alla costruzione di muri e barriere di filo spinato deve essere l'impegno ad avviare progetti di accoglienza integrata non finalizzata unicamente all'assistenza immediata, ma ma all'integrazione sociale ed economica dei richiedenti, al fine di consentire una riconquista dell'indipendenza secondo percorsi personalizzati. Infine, occorre una battaglia di informazione culturale sulla verità contro le bugie e i luoghi comuni. E utilizzo al riguardo le le considerazioni messe nero su bianco da Emma Bonino - non ricordo in questa sede le competenze e la sapienza del personaggio, che è stato vice Presidente del Senato, parlamentare europeo e Ministro

pochissimi (circa 35 milioni) sono gli immigrati, i quali rappresentano una percentuale scarsissima. Paradossalmente, proprio i Paesi più contrari sono quelli che ne hanno di meno. «Non c'è lavoro neanche per gli italiani. Non possiamo quindi accoglierli»: altro falso,

in altissima percentuale, dagli italiani, soprattutto nei settori della cura alle persone, dell'edilizia e dell'agricoltura,

oltre che un impegno concreto su un'iniziativa legislativa corrispondente a una vicenda epocale del nostro Paese e del mondo.

che guardano all'immigrazione come fattore emergenziale, cresce nel Parlamento della Repubblica la consapevolezza di trovarsi di fronte a un fenomeno globale, destinato a durare nel tempo, alimentato da fatti e fattori demografici che certamente mettono addirittura in crisi un concetto che pure è stato finora fondamentale nell'elaborazione della normativa nazionale ed europea, vale a dire la distinzione fra migranti che scappano dalla fame, dalla siccità e dalla povertà e migranti che invece hanno tutti i requisiti per essere considerati titolari del diritto d'asilo o comunque di una protezione internazionale. Cresce altresì la consapevolezza che, a fronte della crescita demografica, l'impoverimento in termini di popolazione dell'Europa necessiterà nei prossimi decenni di avere, a fronte anche dell'invecchiamento della popolazione, la possibilità grazie.

sufficientemente sintetica e orientata a quella che oggi sembra la questione principale, e cioè innanzitutto una questione europea. Non c'è dubbio che il fenomeno della migrazione, che ha impattato così violentemente sui sistemi nazionali, ha impattato con uguale forza, moltiplicata dalle condizioni politiche dei singoli Paesi europei, con una capacità disgregatrice sulla quale si è soffermato il collega Mazzoni. il collega Mazzoni. Per chi è attento alle questioni che riguardano - ad esempio - l'attuazione dell'agenda europea, il dato che francamente si apprezza di più è, da una parte, uno sforzo legislativo e regolatorio dell'Unione europea, che si concreta in una quantità

tutto questo appare come un agire su un piano formale che non riesce a cogliere la natura e la qualità non solo del fenomeno, ma anche della risposta. il senatore Mazzoni, oltre a risultare del tutto inutile, è l'emblema più inquietante di un'Europa che fallisce esattamente su quel piano dell'unità dei valori e dei fini sul quale è stata pensata e costruita. Gli impegni secchi secchi - a nostro avviso - tra le moltissime questioni da affrontare (molte delle quali sono state raccolte nelle mozioni degli altri Gruppi) colgono le misure che il Governo deve assumere in questo momento particolarmente

a quella che è stata una positiva e interessantissima introduzione di tema da parte del Governo italiano, con la lettera informale avente

la Commissione si sta attivando nella confezione delle *fiche* che riguardano i Paesi di provenienza dei flussi migratori, ai quali potrebbero essere riservati accordi di partenariato e forme di finanziamento da grazie. che ogni accordo di partenariato economico e ogni forma di finanziamento non possono prescindere dall'accertamento di alcune precondizioni.

a fenomeni particolarmente gravi e diffusi quali la corruzione che, purtroppo, connotano i Governi di alcuni di essi. infine, altre pochissime considerazioni. Credo non vi possa essere alcuna politica di aiuto nei confronti dei Paesi da cui il flusso migratorio proviene che veda un rapporto esclusivo con i Governi e non coinvolga le forze,

Infine, aggiungo gli altri punti, che mi limito a citare. La mozione in esame conviene con quelle presentate da altri colleghi sulla necessità di sviluppare una nuova politica europea sulla migrazione legale, riesaminando la direttiva sull'ingresso e sul soggiorno per ragioni di lavoro e sulla necessità di intensificare la lotta alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani. Vorrei qui sottolineare che il permanere nel nostro ordinamento della norma sulla

alla piena sicurezza dei cittadini con l'assicurazione della pacifica convivenza civile e dell'osservanza delle leggi. Signora Presidente, abbiamo avvertito l'esigenza di presentare una mozione che prenda spunto da due diversi elementi.

con un atteggiamento, nei confronti della comunità europea, che riteniamo assolutamente sbagliato perché è di natura risarcitoria dal punto di vista economico? No, signora Presidente, è assolutamente sbagliato assumere un tale atteggiamento rispetto a dati che ci dicono esattamente in quale dimensione si prospetta il fenomeno: oltre il 50 per

molto pietosa. Ci vuole un atteggiamento che sia di carattere economico-sociale. Approntiamo uffici immigrazione nei Paesi di provenienza. Tra l'altro, il Senegal e la Nigeria sono i Paesi da cui partono il maggior numero di immigrati. Affrontiamo il problema come se fosse di casa nostra, approntando gli strumenti che abbiamo collaudato in casa nostra.

che non hanno completato il loro viaggio della speranza e in queste ore, mentre noi stiamo parlando, di fronte al mare di Ragusa altri cadaveri vengono recuperati in una situazione veramente tragica. Perché non approntare gli strumenti che conosciamo come civiltà, come popolo europeo rispetto a fenomeni di siffatto genere? Dovremmo non solo conoscere le opportunità

presso i luoghi di partenza, capace di dare le esatte informazioni su dove possono trovare certe risposte e quel minimo di formazione, anche di carattere linguistico, per poter approdare da

Andate in Europa soltanto per chiedere di poter sforare il bilancio dello zero virgola, in virtù delle spese che abbiamo. Sì, questo è un aspetto del problema, ma non è il più importante.

far crescere una nuova cultura capace di alimentare nuove visioni politiche che l'Europa deve saper pronunciare. E dico questo anche quando il contributo offerto si traduce in proposte di impegno rispetto alle quali pronuncerò una posizione contraria da parte del Governo. Come è noto, il Governo italiano ha affrontato il tema dei flussi migratori, che con caratteristiche e andamenti diversi ha interessato il nostro Paese negli ultimi tre anni, cercando sempre di coniugare le istanze derivanti dal diritto internazionale, dalla normativa comunitaria e dalla Costituzione che impongono di offrire accoglienza, con quelle espresse dalla comunità nazionale, che avverte nella pressione migratoria una minaccia alla propria sicurezza e un'insidia alla propria identità. Noi affermiamo ancora una volta come prioritaria la tutela dei diritti e della sicurezza per i cittadini italiani e l'azione tesa a pretendere, da parte degli ospiti, il rispetto delle nostre regole. Siamo convinti che la strada intrapresa sia l'unica capace di far convivere queste istanze, investendo sulle politiche di integrazione e di inclusione e preservando le sacrosante aspettative di sicurezza che esprimono i cittadini italiani. Tanto abbiamo fatto di fronte alla più grande ondata migratoria che l'Italia abbia mai subito: con la straordinaria e proficua esperienza di Mare nostrum siamo infatti riusciti a far accogliere la nostra richiesta che sia l'Unione europea a scendere in mare e a presidiare la frontiera del Mediterraneo.

che l'Unione europea ha proposto attraverso l'agenzia Frontex. Mi riferisco alla più grande operazione di controllo delle frontiere esterne messa in campo dall'Unione europea e realizzata da tale agenzia, che ha l'obiettivo principale di contrastare l'immigrazione irregolare e le attività di traffico degli esseri umani. La visione italiana di una dimensione europea nella gestione del fenomeno migratorio è stata poi fatta propria dalla cosiddetta agenda Juncker, adottata a seguito di un consiglio straordinario dei Capi di Stato e di Governo europei, chiesto e ottenuto proprio dal Governo italiano. La comunicazione della Commissione europea, che va sotto il nome di agenda Juncker, è un documento di grande respiro, sebbene - come è a tutti noto - su alcuni dei suoi punti gravino ancora i condizionamenti e i freni imposti dalle logiche nazionali. È indubbio, comunque, che si tratti di un netto passo in avanti e, soprattutto, di una presa d'atto del cambiamento profondo della realtà migratoria, avvenuto in virtù non di fatti contingenti e di elementi transitori e reversibili, ma dell'azione di fattori di fondo, strutturali, storici e sociali, che chiamano in gioco le scaturigini stesse del fenomeno e che interpellano l'Occidente e l'Europa in una maniera che non era mai stata tanto radicale e drammatica. L'attuazione di tale piano richiede la solidità e l'interconnessione tra i due pilastri di questa nuova politica: la ricollocazione dei migranti che hanno diritto a rimanere in Europa e il rimpatrio di coloro che non ne hanno titolo. Il punto di collegamento tra questi due fondamenti è rappresentato dagli *hotspot*, alla cui creazione l'Italia ha aderito con impegno e determinazione, giungendo addirittura a proporre la creazione di *hotspot* galleggianti o di *hotspot* nei Paesi da cui si originano i flussi. La Commissione europea ha espresso forte apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Italia nell'attivazione di queste strutture, per la straordinaria attività di prima accoglienza che è stata garantita e per il rispetto delle disposizioni europee sul fotosegnalamento, in adempimento dell'obbligo di alimentare il sistema Eurodac. Nell'ambito delle azioni imposte dal piano europeo, il Governo italiano ha realizzato un deciso potenziamento delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale, finalizzato anche al loro trattamento più rapido. Non va dimenticato che l'Italia ha formulato proprie valutazioni sulla proposta di riforma del sistema di Dublino. E la nostra proposta è stata segnalata alla Commissione europea in maniera ufficiale, manifestando in tal modo le nostre fondate riserve sul mantenimento della responsabilità in capo allo Stato membro di primo ingresso e sottolineando al contempo la necessità di dare più spazio al principio di solidarietà. A fronte dei rigurgiti nazionalistici che hanno portato sovente all'inconcludenza dei tavoli europei, l'Italia ha assunto posizioni nette ed espresso posizioni costruttive. costruttive. Come è stato ricordato nei diversi interventi e da ultimo dalla presidente Finocchiaro, anche in ragione del fecondo contributo che quella Commissione ha offerto approfondendo le caratteristiche fondamentali del problema, le tre direttrici vanno gestite perché si possa investire in Africa, si possano risolvere le crisi come quella siriana e le situazioni politiche complesse come quella libica e si possa condividere la gestione dei flussi migratori a livello europeo, evitando di scaricare il peso sui singoli Paesi membri, soprattutto su quelli che sono frontiera esterna dell'Unione. Tale politica - come è noto è stata compendiata nel *migration compact*, che è la proposta italiana diffusa in ambito europeo che ha alimentato un positivo dibattito e segnato alcuni primi risultati, pur tra molte difficoltà. Un passo in avanti in Europa è stato fatto con l'approvazione, recentemente avvenuta, del primo progetto per l'Africa che riprende esplicitamente il *migration compact*. C'è bisogno, però, di un impegno e di una determinazione se vogliamo salvare l'Africa dall'emigrazione e dall'ulteriore impoverimento e l'Europa dalla paura. Dal canto suo, l'Italia prosegue con successo nella sua attività negoziale per rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'area subsahariana. L'Italia può essere il motore di una strategia europea sulle migrazioni, forte di un impegno riconosciuto nei salvataggi in mare, nell'accoglienza di tante persone in difficoltà e nella costruzione di un modello d'integrazione tra culture. In linea con tale impegno, la *governance* nazionale della gestione del fenomeno migratorio si sostanzia anche di un impegno costante nella lotta alle organizzazioni criminali dedite allo sfruttamento dei migranti e alla valorizzazione di tutte le esperienze positive realizzate dalla società civile. Noi esprimiamo un giudizio estremamente positivo per progetti che si stanno realizzando in maniera sostanziale e che vedono direttamente impegnati soggetti della espressione diretta della società civile. Mi riferisco ai corridoi umanitari e alla loro straordinaria valenza di buona pratica e anche di capacità di attivazione di energie nuove e di visioni innovative nell'affrontare questo tema. Il rafforzamento della *partnership* con il mondo delle autonomie locali, introdotta con l'accordo tra Stato, Regioni ed enti locali nel luglio 2014, per la distribuzione sostenibile dei migranti

sul primo impegno il parere è contrario. Sul secondo impegno il parere è favorevole a condizione che venga riformulato con le seguenti parole:

nell'ambito dell'Unione europea di misure urgenti per una gestione più efficace dei flussi migratori, anche mediante l'istituzione di Centri di assistenza nei Paesi del Nord Africa per provvedere in quei luoghi, nel pieno rispetto dei diritti umani e in stretta collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, al supporto e orientamento dei migranti e ai rimpatri volontari assistiti;». Sul terzo e sul quarto impegno il parere è favorevole. Sul quinto impegno il parere è favorevole a condizione che vengano espunte le parole

esprimo parere favorevole a condizione che la parola «ripristinare» venga sostituita con la parola «mantenere» sia espunto il periodo che va dalle parole «anche valutando la selezione dei flussi» fino alla fine.

«a valutare l'opportunità che l'Italia, come Stato membro, sottoponga all'Organizzazione mondiale della Sanità la possibilità di rivedere il Regolamento sanitario internazionale ove se ne ravvisi l'esigenza».

ci fosse però la volontà da parte dei proponenti di rivedere gli impegni che si chiedono in relazione all'applicazione delle norme oggi esistenti, che servono a contrastare anche il fenomeno di illegalità e di spazio per la criminalità organizzata attraverso processi di clandestinizzazione di immigrati, il parere può essere rivisto. In buona sostanza, l'iscrizione all'anagrafe può essere gestita con percorsi più congrui rispetto alle fattispecie trattate e il documento di identità può essere reso efficace per un tempo compatibile con quelli propri della valutazione delle istanze di protezione internazionale.

la riflessione sulla clandestinità fatta dal vice ministro Bubbico su dei punti che toccano la questione dell'iscrizione all'anagrafe comunale e il conseguente rilascio della carta d'identità.

Vogliamo o no sgravare i Comuni dalla nuova incombenza, come anche il prefetto Morcone ha sottolineato la scorsa settimana? Se la risposta del Governo è negativa vuol dire che pone pone un ulteriore aggravio alle amministrazioni comunali e ai sindaci. E di questo noi, come Gruppo della Lega Nord, prendiamo atto.

e che ha orientato il Parlamento, nel varare la legge cosiddetta Bossi-Fini, a definire modalità perché gli immigrati presenti in Italia possano essere identificati e riconoscibili.

favorevole a condizione che vengano sostituite le parole: «a ridurre ai 30 giorni previsti per legge, o comunque in periodi più limitati rispetto a quelli attuali» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di adottare misure anche normative volte a ridurre». Sull'ottavo impegno il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «a promuovere iniziative per una equilibrata distribuzione dei migranti per classe, distribuendo con omogeneità i flussi delle iscrizioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1999».

"«a valutare la possibilità, compatibilmente con le peculiarità dell'ordinamento giuridico italiano di» utilizzare...".

tredicesimo impegno il parere è favorevole, purché venga sostituita la parola «verificare» con la parola «promuovere».

dalle seguenti: «mediante la piena applicazione delle clausole di salvaguardia del regolamento (UE) n.

a porre il tema dell'asilo e dei rifugiati al centro del dibattito europeo, rilanciando la necessità di abolire il regolamento Dublino

il seguente periodo: «l'inserimento di "clausole sociali" da parte delle prefetture in quanto enti appaltanti, atte ad assicurare la continuità occupazionale dei suddetti operatori in occasione dell'avvicendamento delle imprese appaltatrici».

per ricerca di occupazione"; il progressivo trasferimento agli enti locali delle competenze per i rinnovi dei permessi di soggiorno e per l'ottenimento della carta di soggiorno,

un disegno di legge collegato alla legge di stabilità del trascorso anno, che avrebbe dovuto essere esaminato da molto tempo.

la fase complessiva delle dichiarazioni di voto. Il mio Gruppo è quindi senz'altro favorevole a questa sua decisione

Presidente, colleghi, con questo intervento di fine seduta continua oggi, qui al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a quando sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Prego di defluire in silenzio, grazie. Prego, senatrice Capacchione. CAPACCHIONE *(PD)*. Da qualche tempo era tornata dai suoi genitori, non sopportando più minacce e violenze e iniziando il percorso per la separazione.

Nei giorni successivi vi sono stati altri due casi: a Torino, dove è stata uccisa a martellate, per mano del marito poi suicida, Natalina Montanaro, 71 anni; e a Montecerboli, in provincia di Pisa, dove è toccato a Nona Movila, 42 anni, madre di cinque figli, accoltellata mortalmente dal suo compagno, pure lui poi suicida. Salgono così a 21 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. Anche nella Spoon River dell'ultimo fine settimana, però, il femminicidio viene descritto dai giornali come il gesto estremo di uomini disperati, che non riescono ad accettare la separazione dalla moglie o altre comuni avversità, uomini provati dalle difficoltà economiche e depressi. Tutto vero, eppure tutto falso. Le solite spiegazioni di maniera, insomma, che, dando una attenuante al colpevole, addossano alla donna una parte di responsabilità. Il femminicidio invece è quasi sempre 1'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. E lo è anche in questi ultimi casi. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e, nel frattempo, sono stati rafforzati gli strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Stefania, ad esempio, aveva denunciato cinque volte il marito ed era andata via di casa, rifugiandosi dai suoi genitori; ma ciò non è bastato a salvarle la vita. Cosa non ha funzionato dunque, anche in questi casi, nella rete di protezione? Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza.

alla quale gli organi di stampa ci informano di un crescendo di azioni criminali dietro le quali, purtroppo, ci sono sia la 'ndrangheta che la camorra. La presenza di queste associazioni è ormai accertata da inchieste giudiziarie andate a giudizio, le quali dimostrano come i mafiosi avrebbero messo le radici in questo territorio sia infiltrandosi nella cosa pubblica, sia aggiudicandosi appalti, tanto che l'assessore all'ambiente del Comune di Anzio è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, mentre il vice sindaco, Giorgio Zucchini, sarebbe coinvolto in un'indagine per tangenti finite nelle mani della moglie di un *boss* che si trova in

Signora Presidente, ormai conosciamo le manie di grandezza del *premier* Renzi, che hanno portato lo scorso anno a dare disposizione che si allargasse la flotta dei velivoli di Stato. A fianco dei tanti Falcon e Airbus A319,

(40.000 euro al giorno) e chi di 27 milioni all'anno (70.000 euro al giorno) che gli italiani devono pagare, alla faccia della *spending review*!

in occasione del viaggio presso la corte di Obama della scorsa settimana, il *premier* Renzi, con codazzo al seguito, fosse volato con questo Airbus*,* che invece è rimasto

due airbus, doppio equipaggio e doppio carburante. Ora ci chiediamo: che gioco sta facendo Renzi? Perché ha preso un Airbus costoso,

di finti risparmi per promuovere il sì al *referendum*, dica effettivamente agli italiani degli sprechi che sta accumulando, uno dei quali proprio con l'acquisto di questo Airbus, che rimane inutilmente collocato nell'*hangar* di Fiumicino